calendario dei lavori La seduta di oggi sarà tolta subito dopo gli adempimenti relativi al calendario. Questa settimana proseguirà - ove possibile rispetto al parere della Commissione bilancio - l’esame del disegno di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e saranno discussi i seguenti disegni di legge: domini collettivi; aggregazione del Comune di Torre de’ Busi alla Provincia di Bergamo; distacco del Comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al Friuli-Venezia Giulia; istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. Il calendario prevede inoltre la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul raccordo Stato-Autonomie territoriali. La prossima settimana l’Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni 1[a] e 5[a] sul decreto-legge in materia finanziaria attualmente all’ordine del giorno della Camera dei deputati. Nella seduta antimeridiana di martedì 13 giugno, con eventuale prosieguo nella seduta pomeridiana, saranno discusse le mozioni sulla riforma della politica agricola comune e altre in materia agricola. Il calendario della settimana prevede inoltre i disegni di legge sul codice antimafia, ove concluso dalla Commissione, e il decreto-legge in materia finanziaria. In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 giugno si terrà la chiama per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13. Nella seduta antimeridiana di giovedì 15 giugno sarà avviato l’esame del disegno di legge in materia di cittadinanza. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 dello stesso giorno. Le sedute di martedì 20 giugno saranno interamente dedicate alla discussione delle mozioni a procedimento abbreviato sui vertici Consip e sulla proliferazione delle armi nucleari. Il calendario della settimana prevede inoltre le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno. Nella settimana dal 27 al 29 giugno saranno discussi il decreto-legge sull’obbligo delle vaccinazioni

sulla fornitura di servizi rete Internet e - ove concluso dalla Commissione - sulle disposizioni anticipate di trattamento. Nella seduta antimeridiana di martedì 27 giugno sarà discussa la mozione sulla partecipazione di Taiwan a organizzazioni internazionali. Infine, le richieste di informative del Ministro dell’economia sulle banche popolari venete e del Ministro degli esteri sul summit sui Balcani occidentali in programma a Trieste il prossimo 12 luglio potranno essere svolte in Commissione

Signor Presidente, nel corso della seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, durante la discussione sul disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, in in ragione della mia disabilità e dello stato di tensione creatosi e di alcuni errori nella documentazione che portavo con me ho votato in maniera opposta ai miei intendimenti. Chiedo, di conseguenza, la possibilità di consegnare un testo nel quale sono indicati dettagliatamente gli emendamenti che ho votato in maniera erronea e che sia allegato al Resoconto.

La seduta è tolta